riguardato la questura di Milano nelle giornate del 27 e 28 maggio scorsi. Voglio subito premettere che, nella circostanza che mi accingo ad illustrare, la Polizia di Stato ha ancora una volta confermato le doti di professionalità e di equilibrio del proprio personale, che ha applicato con assoluta correttezza tutte le procedure di legge. ore 18,15 del 27 maggio una volante del commissariato di pubblica sicurezza Monforte-Vittoria di Milano interveniva in corso Buenos Aires n. 23 su richiesta di una donna che aveva segnalato di aver subito un furto di circa 3.000 euro di cui, a suo giudizio, era responsabile una sua ospite presente in quel momento nel centro estetico ivi ubicato, che pertanto veniva accompagnata in questura. In base alle procedure ormai consolidate, stanti anche le indicazioni fornite in merito dal pubblico ministero di turno presso il tribunale per i minorenni, venivano svolti tutto gli accertamenti atti all'identificazione della ragazza, che risultava essere Karima el Mahroug, nata in Marocco il 1° novembre 1992 e domiciliata a Milano. Nel corso degli accertamenti, emergeva che la ragazza era da rintracciare perché allontanatasi da una comunità di Messina. La stessa veniva fotosegnalata e, successivamente, compiutamente identificata, anche sulla base delle notizie acquisite dalla questura di Messina e dai genitori della stessa presenti a Letojanni, in provincia di Messina. Tutto ciò avveniva prima della telefonata che, successivamente, alle ore 23 circa dello stesso giorno, il capo di gabinetto della questura di Milano riceveva sul proprio cellulare di servizio da parte di uno dei responsabili del dispositivo di sicurezza del Presidente del Consiglio, che gli passava poi al telefono il Presidente stesso. Riferisce il capo di gabinetto della questura che, nel corso della telefonata, il presidente Berlusconi chiedeva informazioni in merito all'accompagnamento presso la questura di una ragazza di origine nordafricana, che gli sarebbe in precedenza stata segnalata come parente del presidente egiziano Mubarak. Il capo di gabinetto contattava immediatamente il funzionario di turno presso la centrale operativa e apprendeva che effettivamente nel tardo pomeriggio era stata controllata e successivamente accompagnata in questura una minore straniera di origine nordafricana, priva di documenti di riconoscimento e successivamente identificata per la minore in argomento. Il capo di gabinetto chiedeva al funzionario di turno informazioni in merito all'accompagnamento della giovane, raccomandandogli che venissero svolti con celerità tutti gli accertamenti previsti dalla legge. Dopo circa un'ora, intorno alle ore 24, l'addetto alla sicurezza del Presidente del Consiglio richiamava di nuovo sul cellulare il capo di gabinetto chiedendo ulteriori chiarimenti sulla vicenda. Gli veniva risposto che gli accertamenti erano ancora in corso, come da indicazioni provenienti dal pubblico ministero del tribunale per i minorenni. Nel frattempo, giungeva in questura il consigliere regionale Nicole Minetti, che riferiva di conoscere la ragazza, assicurando la propria disponibilità a prendersi cura della stessa. Il funzionario di turno e la centrale operativa, sempre in contatto con l'autorità giudiziaria, accertava che al momento non vi erano posti disponibili nelle comunità della zona; pertanto, considerata l'avvenuta identificazione della giovane, nonché il ruolo del consigliere regionale Minetti e il consenso della ragazza, che affermava di conoscere il consigliere regionale, di cui aveva anche il numero telefonico, sulla base delle indicazioni del pubblico ministero di turno presso il tribunale per i minorenni, veniva redatto il verbale di affidamento. Alle ore 2 del giorno 28 maggio, e quindi circa otto ore dopo il rintraccio, la minore, come emerge dal verbale di affidamento, lasciava la questura insieme al consigliere regionale Minetti; di ciò veniva informato il tribunale per i minorenni con la rituale nota di trasmissione degli atti. Nella gestione della vicenda, quindi, non si evidenzia alcuna modalità che possa richiamare frettolosità o superficialità, avendo gli uffici della questura di Milano rispettato tutte le procedure previste dalla legge, dai regolamenti e dalla costante prassi. Sulla vicenda che ho illustrato, la procura della Repubblica di Milano ha sentito, lo scorso 30 ottobre, il capo di gabinetto e il funzionario di turno come persone informate sui fatti; analoga convocazione ha riguardato, il 1° novembre, il dottor Vincenzo Indolfi, questore di Milano all'epoca dei fatti. Sottolineo poi che il 2 novembre, pochi giorni fa, il procuratore capo della procura della Repubblica di Milano, dottor Bruti Liberati, in relazione al comportamento della questura di Milano e dei funzionari ha dichiarato, cito testualmente, che: «La fase conclusiva della procedura di identificazione, fotosegnalazione e affidamento della minore è stata operata in modo corretto. In futuro non ci saranno altri accertamenti. Per quanto riguarda questa fase dell'indagine abbiamo praticamente chiuso». La correttezza dell'operato della questura di Milano nel caso che ho illustrato è stato così confermata anche dall'autorità giudiziaria. Tutti gli atti relativi a quanto ho descritto sono stati, come sempre, ritualmente trasmessi dall'ufficio minori della questura di Milano alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

ringrazio il ministro Maroni per la puntuale illustrazione che credo abbia dato ai fatti la loro esatta dimensione. Quindi, prendiamo atto delle notizie che, peraltro, erano già state ampiamente riportate e che dimostrano come la questura abbia agito con correttezza, come poi la magistratura ha confermato l'assenza di qualsiasi fatto di rilevanza penale. Nessuno ha impedito il normale corso degli eventi, né quella sera né dopo. La ragazza infatti, come risulta dalla lettura dei giornali, nei giorni successivi è stata indirizzata, essendo stata ulteriormente fermata, ad una comunità; quindi, la questura ha potuto agire in ogni occasione secondo le determinazioni del caso. Prima di lanciare accuse, pertanto, si dovrebbe far abbassare il polverone: si separino verità e menzogne. Mi è capitato di leggere in questi giorni drammatiche testimonianze di madri che hanno sconfessato i deliri delle proprie figlie, smentendo racconti dettati talvolta da autentiche mitomanie di protagonismo. Una delle persone erette a fonte di verità

non si crede a chi racconta di eventi dove nulla è accaduto di ciò che taluni, dando spazio alla fantasia, hanno raccontato? Si crede o non si crede a seconda della convenienza. C'è chi, negli anni passati, annunciava scosse in una singolare sincronia anticipatrice con qualche magistrato. Forse per coprire scandali - quelli sì veri - altamente dannosi per le casse pubbliche - ad esempio, nel caso della sanità pugliese - che hanno visto protagonisti esponenti di una certa corrente politica della sinistra. Né voglio sciorinare scandali e vicende che - come tutti ben ricordiamo - hanno portato alcune Regioni della nostra Nazione al collasso. Chissà cosa scopriremmo se microfoni ed obiettivi, spesso usati in modo illegale, andassero a seguito di tanti personaggi. In questi anni abbiamo avuto banalità elevate a scandalo e scandali ridotti a banalità: c'è chi specula con soldi pubblici, e viene protetto da toghe ed organi di informazione amici, e c'è chi è nemico da colpire per definizione, e quindi da lapidare a prescindere dalla mancanza di responsabilità. In questi giorni abbiamo dovuto sorbirci prediche di ex Ministri della famiglia passati alla storia per avere proposte i Dico; vorrei citare un importante vescovo che nei giorni scorsi ha scritto: «Tra un partito che contemplasse nel suo programma la difesa della famiglia fondata sul matrimonio, e il cui segretario fosse separato dalla moglie, e un partito che contemplasse nel programma il riconoscimento delle coppie di fatto, il cui segretario fosse regolarmente sposato, la preferenza andrebbe al primo partito». Io credo che il centrodestra, quando è stato all'opposizione, abbia avuto il merito di impedire che l'istituto della famiglia venisse svilito e destabilizzato. Il centrodestra al Governo, con Silvio Berlusconi, ha varato provvedimenti di grande importanza per salvare vite umane. Il centrodestra ha difeso e difende la libertà educativa,

la famiglia e, con il centrodestra al Governo, parole come padre, madre, moglie e marito non scompariranno mai dal lessico delle nostre leggi e della nostra società. È difficile, cari amici, subire processi morali da parte di chi propone liberalizzazione di droghe e libertà assoluta per l'immigrazione (anche clandestina), favorendo così il rischio di sfruttamento di donne e di minori;

valore. Cari amici e colleghi, non è tollerabile che da un lato si consideri la sfera privata così sacra e inviolabile da ritenere, ad esempio, che l'autodeterminazione debba

Quando invece la riservatezza viene violata in altri ambiti, bisogna scandagliare, fotografare e radiografare tutto. Noi allora siamo pronti ad accettare anche la sfida della coerenza, su scelte di valori, che voi non siete in grado di portare avanti. E sappiamo bene, cari colleghi, e lo sanno gli italiani, che tutto ciò che accade e che riguarda personalità con ruoli pubblici determina giudizi e valutazioni dei cittadini. Ma, appunto, ciò che accade, non ciò che non accade e che in questi giorni è stato descritto al di fuori della realtà, con falsità che troppi organi di informazione hanno divulgato, scambiando barzellette per realtà e realtà per barzellette. C'era un tempo della doppia morale, in cui, per alcuni tipi di vicende, erano comunque colpevoli alcuni ed altri erano innocenti per definizione; alcuni a sinistra infrangevano leggi ed etica pubblica, ma chi pensava a carriere politiche con la sinistra chiudeva gli occhi, pur indossando una toga o dirigendo organi di informazione. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Per alcuni il mondo va così, con la logica della doppia morale, che noi vogliamo denunciare senza tacere della vostra ipocrisia.

degli stili di vita personali e, soprattutto, delle proposte politiche a tutela della vita, della persona e della famiglia, non prenderemo mai lezioni da chi vuole devastare questi valori e questi principi, che il Popolo della Libertà difende sempre e comunque.

ministro Maroni, lei ha tenuto a precisare al Parlamento che i funzionari e gli agenti della questura di Milano, quella famosa notte tra il 27 e il 28 si sono comportati in modo assolutamente rigoroso e rispettoso della legge. Noi ne siamo convinti e mi permetta di dirle che il Gruppo del Partito Democratico al Senato manifesta pieno rispetto e piena solidarietà a tutto il personale della questura di Milano.

è che - appunto - quel lavoro serio ed ordinato di un ufficio di Polizia in uno Stato democratico e la serenità di chi svolge un lavoro che ha ad oggetto beni pubblici assai preziosi possono soffrire né limiti, né pressioni, né tempi che non siano quelli dettati esclusivamente dalla più puntuale applicazione della legge. Quel lavoro va rispettato: così, però, non fu quella sera perché quel lavoro venne scandito dall'intervento ripetuto (di cui lei peraltro ha fatto menzione), allarmato, pressante e condito di menzogna del Presidente del Consiglio e di un soggetto delegato, che non poteva essere delegato perché era il suo capo scorta. avveniva mentre la questura di Milano affrontava la questione di una minorenne non italiana, sfuggita all'affidamento operato da un'autorità giudiziaria minorile, e che era denunciata per furto: in tale situazione, il primo interesse della questura di Milano era quello della minore che si trovava con tutta evidenza in una stituazione di vero e serio sbandamento. Evidentemente, e per candida ed espressa ammissione dello stesso presidente Berlusconi, né un ufficio della Polizia di Stato né una comunità di accoglienza per minori sono luogo abbastanza sicuro per una minorenne! Tralascio, per carità di Patria, altri luoghi ed altre occasioni in cui il presidente Berlusconi l'avrebbe tenuta al sicuro (*Applausi dal Gruppo PD*). Per questo, bisognava farla uscire al più presto da quell'ufficio di questura e, per questo, si è abusato di verità e di potere per affidarla ad una persona appositamente inviata lì, nel cuore della notte, che pure riveste pubbliche funzioni ed esercita pubbliche responsabilità, e che era incaricata di lasciarla andare via, cioè di abbandonarla, con il risultato che una settimana dopo quella stessa minorenne verrà aggredita e ricoverata in ospedale, trovata dalla Polizia in casa di una donna brasiliana che, stando alle sue dichiarazioni, voleva indurla alla prostituzione.

È risibile soltanto pensarlo! È stato nell'interesse evidente del Premier, per evitare domande dovute nell'occasione dalla Polizia di Stato che potessero svelare condizioni di vita, abitudini e frequentazioni di una minorenne in vera difficoltà. Perfetto! Ciò che tutti vedono è un Presidente del consiglio che comunica al Paese che una minorenne in un ufficio di questura è in pericolo; un Presidente del Consiglio che è in evidente e irrefrenabile agitazione per le conseguenze che possono derivare da un accertamento di polizia; un Presidente del Consiglio che mente, che abusa del suo potere e che, soprattutto, ancora una volta, pensa solo a se stesso. La vicenda è questa e non c'è molto altro da dire. Anche su tale piano - e lo ripeto - Silvio Berlusconi si conferma inadeguato ad essere il Presidente del Consiglio di un grande Paese democratico! PD*). Rumoreggiate, non potete dirlo, ma molti di voi sono consapevoli di questo; lo è certamente quel pezzo dell'originaria maggioranza, consistente a sufficienza per essere determinante ai fini di un'eventuale fiducia alla Camera dei deputati, che si raccoglie intorno al presidente Fini. Voi non ne volete sentire parlare, invece bisognerà parlarne perché il Paese non è più in grado di sopportare e perché il rischio che si apre per l'Italia è quello della palude, mentre incombono responsabilità enormi, alle quali evidentemente sfuggite. Anche solo limitandoci ad una questione (che discuteremo proprio in questi giorni), cioè il piano nazionale delle riforme, vorrei sapere se un Governo che rischia di non poter muovere un passo per la situazione di stallo in cui si è cacciato possa ottemperare all'impegno di ridurre di 45 miliardi di euro il debito.

Può essere questo Governo, con questo Presidente del Consiglio, a rappresentare con autorevolezza il Paese e a presentare autorevoli proposte e presenza in Europa per evitare la marginalizzazione e la totale irrilevanza dell'Italia? Qui emerge l'anomalia del PdL e le conseguenze che ciò comporta sul Governo del Paese. Il Paese sarà costretto al rischio di precipitare perché nel più grande partito italiano, quello che voi rappresentate, colleghi, che ha avuto un credito altissimo di fiducia degli italiani, tra i tanti dirigenti che affollano questi banchi e quelli della Camera e le più alte e prestigiose cariche all'interno del partito, non circola e non ha ospitalità il principio di responsabilità nei confronti dell'Italia. In un Paese normale, in un partito normale, l'anomalia e l'inadeguatezza di questo Presidente del Consiglio sarebbe stata ovviata e risolta, con ogni riguardo naturalmente, in nome della responsabilità che avete nei confronti dell'Italia, ma voi non ne siete capaci. È questo che vi manca. Troppo leaderismo, troppo fanatismo, troppo *porcellum*, troppo «meno male che Silvio c'è», hanno fatto di voi dirigenti politici portavoce senza più voce, e questo mentre Bossi lancia l'OPA sul Governo, un Governo sempre meno a marchio PdL e sempre più a marchio Lega. Di ciò dovremo tornare a parlare e vi giuro che lo faremo.

*(LNP)*. Signor Presidente, ministro Maroni, rappresentanti del Governo, colleghi, prendiamo atto ancora una volta che l'unica cosa che sanno fare le opposizioni è alimentare inutili polemiche che non servono al Paese e che vanno ad avvelenare ancora di più, se possibile, il clima politico. Prendiamo atto ancora una volta che in questa legislatura, senatrice Finocchiaro e cari colleghi del centrosinistra, avete deciso di specializzarvi nella politica del *gossip*. L'abbiamo visto con il caso D'Addario. Per un anno intero avete parlato solo di quello, sperando così di indebolire il Governo e guadagnare consensi. Così non è stato e alle ultime elezioni regionali avete subito l'ennesima clamorosa sconfitta. Una lezione però che non vi è servita, tenuto conto delle dichiarazioni degli ultimi giorni. Il Ministro, che ringraziamo per la puntuale informativa, è stato molto chiaro. La questura di Milano ha rispettato tutte le procedure di legge riguardo al rilascio della ragazza in questione. Nessuna irregolarità, nessun favoritismo. Le telefonate arrivate da palazzo Chigi non hanno in alcun modo interferito, né corretto l'operato della questura. Tutto ciò, era comunque già noto a tutti ed è stato confermato nei giorni scorsi anche dalla procura di Milano. E allora, perché questa informativa? Perché chiedere al Governo di riferire in Aula su una questione già ampiamente chiarita? Perché invece di discutere di problemi seri, dei veri problemi del Paese, siamo costretti oggi a perdere tempo su questo argomento? Lo stiamo facendo - è giusto ricordarlo a chi ci sta guardando da casa - per volontà delle opposizioni. I Capigruppo del centrosinistra non hanno chiesto un dibattito in diretta televisiva sui problemi collegati alle devastanti alluvioni che hanno colpito negli ultimi giorni diverse aree del Paese. hanno voluto e preteso questo dibattito semplicemente per sparare ad alzo zero contro il Governo. Siamo, cari colleghi, l'unico Paese al mondo in cui le opposizioni passano il loro tempo a guardare dentro il buco della serratura della casa dei loro avversari politici. Questa la verità. ognuno è libero di fare quel che crede, anche di continuare a sbagliare. Dico solo che, per quanto ci riguarda, il caso Ruby, chiamiamolo così, c'interessa poco. La Lega Nord non parteciperà al dibattito in corso sui giornali e le televisioni; preferiamo dedicare il nostro tempo ad altro e ai veri problemi del Paese. E visto che ne abbiamo l'occasione vogliamo ringraziare il ministro Maroni per l'ultimo pacchetto sicurezza che ha presentato la settimana scorsa in Consiglio dei ministri Nonostante le polemiche - e ce ne sono davvero tante in questi giorni - gli uomini della Lega continuano a lavorare nell'interesse dei cittadini e del Paese. Dopo il successo del primo pacchetto sicurezza voluto dal nostro Ministro, che è riuscito a bloccare i flussi dei clandestini in arrivo nel nostro Paese e che ha portato una notevole diminuzione dei reati cosiddetti comuni nelle nostre città, con il secondo pacchetto si va a completare il programma elettorale presentato agli elettori nel campo del contrasto alla criminalità. Così, mentre voi in Aula, cari colleghi delle opposizioni, parlate di veline, noi diamo più poteri ai nostri sindaci per il controllo del territorio mentre voi vi occupate di festini, noi investiamo al meglio gli ingenti beni confiscati alle cosche mafiose per destinarli alle forze dell'ordine e mentre voi vi occupate di *gossip,* noi provvediamo a regolare l'espulsione dei cittadini comunitari che non hanno diritto a restare sul nostro territorio. Mi spiego meglio. I rom e gli zingari che sono entrati nel nostro Paese, provenienti dalla Romania o da altri Paesi dell'Europa dell'Est, che sono venuti a casa nostra senza nessuna intenzione di integrarsi

Chi si integra, lavora e paga le tasse può rimanere. Chi invece di lavorare ruba, chi invece di integrarsi decide di sfruttare i propri figli nell'accattonaggio, facendoli vivere nel degrado e in mezzo ai topi non è il benvenuto e deve essere espulso. Queste, colleghi, sono le risposte che dà la Lega: sicurezza nelle città, a casa propria e nelle nostre strade. Questa è la politica del fare, non la politica delle chiacchiere che state portando avanti voi in Parlamento. E visto che ne abbiamo l'occasione, vogliamo ringraziare il ministro Maroni anche per i grandi successi che sta ottenendo nella battaglia contro la mafia. Risultati mai visti prima:

Un provvedimento per rilanciare l'economia del Mezzogiorno. Ma tutto questo sarà possibile perché le aree interessate sono state preventivamente bonificate dalla criminalità. Lo sradicamento della criminalità organizzata è l'unica precondizione per garantire sviluppo e progresso e per far radicare su quei territori la cultura del lavoro che ha fatto del Nord il motore economico del nostro Paese. Continueremo, signor Presidente, con la politica del fare: al Governo coi nostri Ministri e in Parlamento. Il nostro Gruppo è il più presente al Senato e non certo per strappare un voto alla voce delle presenze; non ci interessa questo. Siamo qui per onorare il mandato elettorale. per dare risposte ai cittadini e continueremo a farlo, cari colleghi delle opposizioni, senza farci condizionare dal *gossip* del giorno e dai giochi e dalle congiure di palazzo. Detto questo, concludo il mio intervento, signor Presidente, ringraziando, anche a nome di tutti i senatori del mio Gruppo, il ministro Bossi e il presidente Berlusconi per essere stati oggi in Veneto tra i nostri alluvionati. La mia terra - sono veneto - è stata devastata da un'alluvione senza precedenti, con migliaia di sfollati, fiumi esondati, città allagate, danni ingenti all'agricoltura e alle imprese.

perché questa è la miglior risposta che si può dare alle migliaia e migliaia di cittadini che stanno soffrendo, che hanno perso tutto e che non capiscono perché nei palazzi della politica e in Parlamento si parla di altro.

vorrei prima di tutto dire a chi ha sottolineato l'esigenza di una diretta per il Veneto che forse è stato meglio così, perché tutta la gente, tutto il popolo italiano avrebbe potuto sentire i ripetuti «Andatevene a casa!» nella contestazione che c'è stata stamani.

sono giorni bui per le nostre istituzioni ma, signor Ministro, ci consola constatare che tra le rare eccezioni al grave quadro di degrado generale spicca il suo Ministero. In tanti la settimana scorsa abbiamo tirato un sospiro di sollievo nel vederla assumere prontamente le difese della Polizia di fronte all'ennesimo scandalo che ha travolto la politica. Inizialmente, infatti, da diverse parti si è tentato di scaricare le colpe e le menzogne del cosiddetto caso Ruby sulle forze dell'ordine, gettando fango su una questura che ho avuto l'onore di dirigere e di cui conosco l'assoluta professionalità.

di Milano, che al pari di tutte le altre in Italia è gravemente penalizzata dalla inadeguatezza delle risorse e dalla continua emorragia di fondi. È eroico, a mio avviso, lo spirito con cui negli ultimi tempi i nostri uomini e le nostre donne in divisa hanno continuato a svolgere il proprio dovere proseguendo la lotta alla criminalità organizzata e completando indagini costate anni di paziente lavoro. Tutto ciò a dispetto dei tagli agli straordinari; tutto ciò a dispetto di mezzi tecnici vetusti e usurati; tutto ciò a dispetto dell'ormai fisiologica carenza di organico e, soprattutto, in barba alle promesse dispensate dal Presidente del Consiglio durante la campagna elettorale: «mai, mai, mai», si disse in più occasioni, «taglieremo risorse alle forze dell'ordine». Non solo, onorevole Ministro, nonostante i suoi sforzi - di cui ancora una volta voglio dare atto - tale promesse, come tante altre, sono state a più riprese tradite, ma nei giorni scorsi sulla nostra Polizia è piombato anche il peso di una nuova beffa, la beffa, appunto, della vicenda Ruby. A proposito, signor Ministro, sarà bene poi sapere che fino farà questa Ruby, dai Gruppi PdL e LNP)*. Fortunatamente la magistratura, quella magistratura tanto vituperata che ancora oggi è stata offesa e insultata in modo generalizzato, ha subito accertato la correttezza delle procedure seguite dalla questura. Non voglio tornare sui particolari di quella notte e di quelle telefonate giunte dall'alto; ma voglio chiedermi, questo sì, se il presidente Berlusconi, che ha giustificato il proprio intervento presso la Polizia come un atto di generosità verso una povera sfortunata, si sia mai prodigato allo stesso modo e con tanto interesse per altri sfortunati, spinti ad azioni illecite dalla malasorte e dalla inesperienza della giovane età. E sì che in Italia, e nelle questure in particolare, onorevole Ministro, di simili sfortunati se ne contano in abbondanza. Rinunciamo, tuttavia, a questa risposta e guardiamo oltre. Sebbene infatti il Paese sia stufo di continui scandali e sebbene sia innegabile il peso e l'interesse pubblico della vita privata di un Presidente, noi siamo oggi pronti a minimizzare l'accaduto. Hanno ragione quanti nella maggioranza sostengono che non si possa per il caso Ruby far cadere un Governo. Né le presunte denunce delle scorte presidenziali, usate per scopi decisamente impropri;

Tutto ciò ci interessa, ci indigna e ci sconforta, ma vale poco a fronte dei drammatici problemi sociali ed economici che stanno affliggendo il Paese reale, laddove il tasso di disoccupazione continua a salire, i giovani sono paralizzati da una precarietà dilagante e la scuola e l'università da troppo tempo non sono più all'altezza della loro missione civile e sociale. a imporre le dimissioni del Governo dovrebbe essere questa semplice evidenza: l'evidenza del suo fallimento politico. Non solo, infatti, le promesse elettorali di tre anni fa sono state tradite, ma lo stesso programma in cinque punti riproposto al Parlamento a fine settembre come agenda da realizzare in quattro settimane è rimasto lettera morta, ad esclusione - naturalmente - del capitolo federalismo: un tributo alla Lega che poco incide sul malessere dilagante del Paese. Nulla di fatto, dunque, e nessuna assunzione di responsabilità, perché la colpa dell'incapacità e dei gravi ritardi del Governo viene sempre trasferita altrove: sui magistrati, sulla stampa, sui comunisti in genere. Questa etichetta viene brandita come una clave sull'opinione pubblica. Dunque, onorevole Ministro, tramite Ministro, tramite la sua stimabile persona vorremmo far oggi arrivare al Presidente questo messaggio: l'Italia langue in uno stato di grande sofferenza e il Premier, in virtù della sensibilità, della moralità e dell'attaccamento al Paese che ha sempre sostenuto di avere, dovrebbe oggi farsi da parte. Lasci ad altri l'arduo compito di inaugurare una nuova stagione politica, dove i rappresentanti eletti dal popolo possano concentrarsi esclusivamente sui problemi della società e sulle soluzioni possibili. Il suo tempo è scaduto. finestra") *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, lei ci garantisce che che nella questura di Milano sono state seguite nel modo più preciso le procedure. Noi siamo molto contenti di ciò, perché eravamo preoccupati per i funzionari della questura, che avrebbero potuto essere incolpati di atti irregolari. Permarrebbero dei dubbi, per la verità. Le case famiglia disposte ad accogliere la ragazza pare che fossero almeno quattro l'affidamento a un consigliere regionale, che si qualifica consigliere regionale con incarico alla Presidenza del Consiglio (incarico misteriosissimo), lascia qualche dubbio. purtroppo, sappiamo che l'affidataria ha lasciato la ragazza a una persona brasiliana, che qualche giorno dopo pare abbia anche provato a prostituirla, ma questo non tocca l'operato della questura. Siamo sollevati per la regolarità che il Ministro ci garantisce, per un motivo fondamentale:

Rilevo di passaggio che il comportamento regolare della Polizia ha quasi subito accertato la menzogna sull'identità della ragazza, perché si è scoperto che la sua identità era un'altra. quindi è sotto l'attenzione pubblica oggi, cari colleghi e signor Ministro, non è l'operato della questura, bensì la gravissima telefonata del Presidente del Consiglio, allertato non si sa bene da chi: da persona che, chissà perché, disponeva del suo cellulare e che ha suscitato in lui una grave preoccupazione. Si è trattato di una preoccupazione così grave da spingerlo a impersonare un ruolo degno di una farsaccia di Totò. Perché sostenere che la ragazza è la nipote di Mubarak è una menzogna grossolana, ridicola ed imbarazzante anche per le nostre relazioni internazionali. Tra l'altro, forse il Presidente del Consiglio non sa che la distanza tra il Marocco e l'Egitto è grosso modo quella tra la Calabria e la Danimarca. Ma l'elemento fondamentale della menzogna del Presidente del Consiglio è che la richiesta del rilascio - e questo sta agli atti e lo si può ricostruire - previene la procedura d'identificazione e questo specifico atto poteva costringere i poliziotti della questura di Milano a compiere una grave irregolarità.

da una provvidenziale amnistia; ha mentito sulla famosa All Iberian, giurando persino sulla testa dei suoi figli, (che in virtù di questi atti rischiano di perdere la testa un giorno o l'altro) sul non possesso della suddetta azienda, che è invece la cassaforte delle procedure di corruzione della magistratura. Mentitore abituale! L'aspetto più importante della menzogna abituale è che in realtà essa si concretizza come un vero e proprio abuso in atti d'ufficio, un abuso di potere un abuso di potere odioso: perché un potere sovrastante che influisce in modo insinuante ed ipocrita su funzionari pubblici, inducendoli a commettere delle irregolarità, è un abuso di cui

Purtroppo devo rilevare, signor Ministro, che anche il capo del suo partito ha avuto un'indulgenza nei confronti di questo atteggiamento; perché quando Bossi ha dichiarato, in modo del tutto sconvolgente, che sarebbe stato meglio se Berlusconi avesse chiamato lui oppure lei, signor Ministro il capo del suo partito, senza rendersene conto, (forse cercando di mettere una toppa peggiore del buco) ha rivelato anch'egli una concezione privatistica del potere, come se un problema di questo tipo fosse risolvibile semplicemente tramite un patto privato tra persone. Qui si parla della cosa pubblica e dell'interesse collettivo, non di faccende che possono essere risolte con telefonate tra persone private, interessate a un fattaccio privato e ad una farsaccia privata. In conclusione, la menzogna e l'abuso di potere

Chi si comporta in questo modo non ha diritto neanche di pensare di poter salire al soglio maggiore della Repubblica, dove si deve salire con onore, discrezione e capacità di rappresentare bene e al meglio ciò che la Nazione esprime. *(Applausi Chi si è macchiato di questa cosa non solo non può più pensare d'ora in poi di salire al Quirinale, ma non è più nemmeno degno di sedere al posto di Presidente del Consiglio: chi esercita in modo sistematico menzogna ed abuso di potere non può stare a palazzo Chigi. Dimissioni!

Appare davvero singolare ed anomalo, signor Ministro, che nel momento in cui il Paese è alle prese con enormi problemi finanziari, economici e sociali, questo Parlamento debba occuparsi di una vicenda a prima vista di *gossip*, ossia delle notti brave del Presidente del Consiglio. Tuttavia, come ha giustamente osservato il professor Rodotà, la distinzione tra vita privata e vita pubblica, sacrosanta nel caso di cittadini comuni, quando si tratta di un personaggio pubblico di primo piano, non ha molto senso: sul caso sul caso che stiamo discutendo alcune domande dobbiamo porcele. Dalla ricostruzione del presidente Berlusconi pare che non fosse nota la minore età della ragazza e che si fosse preso per buono il suo rapporto di parentela con il presidente Mubarak. Si deve dunque desumere che persone non precisamente identificate entrano ed escono dai palazzi del potere e dalle residenze del Premier? E allora esiste o no, signor Ministro, che riguarda non solo la persona del Presidente del Consiglio e i connessi rischi di condizionamenti e ricatti, ma ancora di più la sicurezza delle istituzioni? E ancora: è normale che per una ragazza extracomunitaria minorenne - e a lei sta molto a cuore, signor Ministro, la problematica degli extracomunitari accusata di furto e di cui non si conosce esattamente l'identità si intervenga presso la questura di Milano facendo pressione per riservarle un trattamento di favore? La stessa giustificazione del Presidente del Consiglio non è condivisibile. Non può essere detto: l'ho fatto perché sono buono, l'ho fatto per bontà, l'ho fatto per aiutare i deboli. Perché in questo caso non bisogna fare privilegi ma bisogna assolutamente aiutare tutti. Guardando al problema da un punto di vista più generale, non si può non rilevare come ci si trovi di fronte ad una situazione di serio degrado dell'etica pubblica. Di questo avremmo dovuto parlare; di questo avrebbe dovuto parlare lei, oltre che raccontarci in maniera chiara la vicenda di quella notte. Se a destra come a sinistra le frequentazioni delle ragazze con uomini potenti sono opportunità per le stesse di raggiungere gli ambiti traguardi di apparizioni televisive e persino di carriere politiche, il modello culturale che emerge da questa vicenda, signori Ministri, la visione della donna è sconvolgente. È sconvolgente quello che abbiamo sentito in questi giorni sulla visione della donna, del suo ruolo nella società, dei parametri,

per questa vicenda. Questa bufera su Berlusconi e sulla sua corte di ragazze sta provocando ondate di reazioni, anche in senso opposto, signor Ministro, che comunque trasmettono un messaggio poco edificante ai giovani. Lo so, nella società di oggi ci sono veramente percezioni

perché il più grande editore gossipparo certamente non sta da questa parte: chi fa soldi con i *gossip* sui giornali, sui settimanali molto noti di cui si vendono milioni di copie, certamente non appartiene alla nostra cultura. Il nostro Paese è cambiato molto in fretta e sicuramente non è stato ininfluente l'ingresso della televisione privata, che fa il suo mestiere e a cui si è progressivamente uniformata anche quella pubblica. Ho ascoltato con qualche perplessità le parole con cui l'onorevole Giovanardi ieri giustificava l'assenza del presidente Berlusconi all'apertura della Conferenza sulla famiglia e ammoniva a non intromettersi nella vita privata dei leader politici, perché pochi di essi ne uscirebbero esenti da colpe. Questo significa che si può tranquillamente professare il più alto ideale della moralità, di attaccamento ai valori della famiglia e della religione e contraddirli poi il giorno dopo. Forse dobbiamo amaramente rimpiangere la cosiddetta prima Repubblica - lo dicono tante persone in questi giorni, non chi lo ha detto nel comizio di domenica - dove l'esempio delle più alte personalità politiche contribuiva alla valorizzazione di un'etica pubblica oggi praticamente inesistente.

Signor Presidente, signor Ministro, signori colleghi, ho riflettuto mentre ascoltavo gli interventi dei colleghi su quale approccio utilizzare per intervenire sulla vicenda e sulle considerazioni, sulla relazione del ministro Maroni: se cioè utilizzare il filo della cronaca. Poi mi sono detto che, nell'epoca del tempo reale la cronaca corre così rapidamente che mentre ne parli è già domani, per cui vi è il rischio di occuparsi del passato oppure di restare in superficie e quindi di essere superficiali, banali, banalizzanti, cinici. Ed allora, forse l'approccio più giusto è quello di considerare l'esemplarità di alcune vicende, perché mi hanno insegnato qualche tempo fa che la politica dovrebbe occuparsi della profondità di quel che accade, accade, recuperare la radicalità delle questioni, dei problemi, delle idee e dei valori, cercare di scandagliare per capire che cosa accade nel profondo di una società. Ed in fondo la vicenda di cui ci stiamo occupando è da questo punto di vista una vicenda esemplare della società italiana, del tempo che viviamo, delle contraddizioni che la società italiana esprime. Signor Ministro, abbiamo accolto con grande favore il fatto che lei abbia avuto l'assetto della sua carica istituzionale nel difendere fino in fondo le forze dell'ordine. Le forze dell'ordine meritano di avere un Ministro che ha questa capacità di decisione e di scelta di campo; ed abbiamo preso atto con soddisfazione che le forze dell'ordine nella vicenda milanese si siano comportate con correttezza e con esemplarità. Eppure è questa la contraddizione, lo specchio di questo Paese. Forze dell'ordine, scarso stipendio, servitori dello Stato discreti, con l'etica e con la cultura del dovere in un Paese, in un contesto metropolitano segnato dal lusso, dal materialismo sfrenato, dall'utilizzo del corpo per fare successo, dalla strada breve che passa attraverso una *lap dance* ed un festino

e la contraddizione di questo Paese e non solo una vicenda istituzionale fin troppo chiara ed evidente. Guardate, ve lo devo dire con grande onestà intellettuale e con grande chiarezza. Sentendo alcune difese del Presidente del Consiglio ho apprezzato la schiettezza, l'onestà intellettuale a suo modo, nel bene e nel male - del presidente Berlusconi, che credo sia il primo a riconoscere gli errori e che anche dal punto di vista dei comportamenti istituzionali quella telefonata non andava fatta rispetto ad un eccesso di zelo che non prende per buone le realtà, i fatti, i comportamenti, non le vicende di carattere penale che non ci riguardano e che non ci interessano. Credo che dobbiamo utilizzare questa vicenda e questa circostanza per affrontare certi problemi e per sciogliere certi nodi. Non è senza significato che il Presidente del Consiglio non abbia aperto il *Forum* delle famiglie e che abbia ritenuto di non intervenire per evitare strumentalizzazioni.

di affrontare i problemi della famiglia italiana e del degrado valoriale cui stiamo assistendo. Per questo credo che tutti insieme dobbiamo esprimere una coralità, al di là della contrapposizione perenne, continua e costante, al di là del rimpallarsi responsabilità, al di là di questa sorta di ping-pong del fango, (che uno butta da una parte e l'altro respinge buttandolo dall'altra parte) perché forse non comprendiamo fino in fondo che ci troviamo in una condizione in cui cui o la politica recupera fino in fondo il suo senso alto, nobile e significativo, o non vince una parte contro l'altra perché c'è una crisi di sistema diffusa e generalizzata che significa la rottura, la lontananza del rapporto tra cittadini e politica, tra cittadini ed istituzioni. Da questo punto di vista tutti, tutti noi, senza la pretesa di essere i primi della classe, dobbiamo chiedere più sobrietà, più capacità di rispettare la funzione pubblica che ci viene attribuita, più capacità di muoversi in una dimensione che recuperi complessivamente l'etica della responsabilità e che restituisca ai cittadini la fiducia nella politica e nelle istituzioni.

ha approvato modifiche e integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 18 novembre. Oggi pomeriggio riprenderanno le votazioni sugli emendamenti e gli articoli del disegno di legge di riforma della professione forense.

Domani mattina alle ore 9,30 sarà posto all'ordine del giorno il progetto di Programma nazionale di riforma, assegnato alla 5a Commissione permanente con le osservazioni di tutte le altre Commissioni. Per 1'esame del documento, cui è abbinato il seguito della mozione Rutelli ed altri sulla politica economica, si è proceduto alla ripartizione dei tempi tra i Gruppi, al fine di concludere le votazioni sugli strumenti di indirizzo entro la fine della seduta antimeridiana di domani per la quale non è previsto l'orario di chiusura. Nella seduta pomeridiana di domani e nella seduta antimeridiana di giovedì prossimo proseguirà la discussione del disegno di legge di riforma della professione forense, domani alle ore 19, il Sottosegretario per la Protezione civile renderà un'informativa sui recenti eventi alluvionali; inoltre, nella mattina di giovedì, alle ore 10,30, il Ministro per i beni e le attività culturali riferirà sul crollo della Casa dei gladiatori a Pompei. Per entrambe le informative sono previsti interventi dei rappresentanti dei Gruppi per 5 minuti ciascuno. Il calendario della settimana corrente prevede inoltre ove possibile in relazione all'andamento dei lavori - la discussione della mozione Ghedini sui benefìci a favore delle vittime del terrorismo e della mozione Li Gotti sulle candidature elettorali. La prossima settimana, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, 1'Assemblea esaminerà una proposta di conflitto di attribuzioni su questione concernente l'*ex* ministro Mastella, nonché il disegno di legge recante esecuzione domiciliare di pene detentive non superiori a un anno, ratifiche di accordi internazionali e la mozione Baio ed altri sulla patologia della depressione. Queste le decisioni che la Conferenza dei Capigruppo ha assunto all'unanimità.

Sono presenti in tribuna gli studenti dell'istituto tecnico «Mattei» di Isernia. A loro rivolgiamo il nostro saluto e gli auguri per la loro attività di studio. punto all'ordine del giorno, che è il seguito della discussione dei disegni di legge sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Colleghi, non si può andare avanti così. Chi deve parlare vada fuori, per favore; non si può procedere così.

conforme al relatore.

**Il Senato non approva**.

conforme al relatore.

perché sia, in qualche modo, garantita la pari rappresentatività negli organismi dell'ordinamento forense. Questa norma mi sembra sia in tendenza e anche rispettosa dei principi costituzionali.

escludere dalla composizione dell'ordine il consiglio istruttore di disciplina e il collegio giudicante. Abbiamo creato un qualcosa che fa, disfa e giudica qualsiasi cosa e se non si dovesse porre un limite anche all'elezione consecutiva - non alla rielezione - (come intende fare anche il senatore Bornacin), si andrebbe in qualche modo modo a creare qualche cosa di molto consolidato, indiscutibile e indiscusso che si potrebbe protrarre negli anni. Non ci sembrava pertanto di essere stati particolare punitivi con questa misura, che, questa misura, che, tra l'altro, è già applicata in altri consigli e consessi elettivi, come il consiglio regionale, al quale noi abbiamo consentito tutta una serie di esclusioni. Ricordo il dibattito che abbiamo svolto relativamente ai consiglieri e assessori regionali. Diciamo che per analogia si riteneva opportuno porre due mandati e la possibilità di ricandidarsi

abbondano disposizioni a tutela dell'interesse degli avvocati, ma fa difetto la parte in cui si tutela in modo preciso, concreto e moderno (che tiene conto delle esperienze più delle esperienze più rilevanti e interessanti che ci offre il panorama internazionale)

tra il cliente e qualsiasi professionista, è l'asimmetria informativa che pone sovente il cliente in una posizione di debolezza e di

Tutti sappiamo, perché fa parte della coscienza diffusa, quanto sia problematica la posizione di una persona che ha

il parere di un altro legale indipendente che se del caso tranquillizzi il cliente sul fatto che l'assistenza che gli è prestata è corretta, che non ci sono conflitti d'interesse e non ci sono errori evidenti nel modo di procedere. Diverse associazioni professionali in altri Paesi offrono proprio questo, ossia la possibilità di avere una *second opinion* riservata e gratuita, a garanzia dell'affidabilità dei membri dell'associazione.

di controllo che può essere adito direttamente in modo riservato, senza conseguenze dirette né per il cliente né per l'avvocato?

cliente. La grave asimmetria informativa che caratterizza il rapporto in questo caso giustificherebbe in modo particolare l'introduzione di una forma Credo che il prestigio dell'avvocatura non avrebbe che da guadagnare dall'introduzione di un servizio di questo tipo. La stragrande maggioranza degli avvocati, che svolgono con coscienza e con perfezione tecnica e professionale il proprio lavoro, non avrebbero nulla di che dolersi dell'esistenza di un servizio di questo genere; mentre l'intera categoria avrebbe il vantaggio di presentarsi al Paese con un elemento di trasparenza e di amichevolezza - possiamo chiamarla così - nei confronti degli utenti del servizio. Oggi chi ha un dubbio sulla correttezza del comportamento del proprio patrono è totalmente indifeso, non ha modo di verificarlo. Correggere tale situazione riporterebbe un po' questa legge a quella che dovrebbe essere la sua funzione, cioè la tutela del cliente. Per questo chiedo che all'emendamento 28.200 il relatore e il Governo prestino particolare attenzione.

della chiusura e della miopia con cui la maggioranza ha affrontato e sta affrontando questo disegno di legge, pure tanto importante.

contenuta, limitata, compressa. Sia chiaro, non vogliamo continuare a dire che non ci basta mai quello che viene concesso, ma la strutturazione dell'istituto, nel modo con cui l'ha determinata, l'ha voluta e l'ha accolta la maggioranza prelude ad un *flop*, ad una non attuazione dell'istituto, che, ripeto, è di grande profilo di civiltà. Perché dico questo? Che vuol dire accettare un istituto come lo sportello per il cittadino e poi scrivere nella legge che l'ordine degli avvocati può istituirlo? Che vuol dire? Vuol dire che alcuni ordini lo istituiranno ed altri no. Ma questo non va bene, perché siamo tutti cittadini di serie A, quelli del Sud, del Centro e del Nord. In tutte le parti del Paese, in tutti i luoghi, in tutti i

Non c'è quindi nessun pericolo: questo lo avete compreso bene e avete accettato l'istituto. Ma è grave prescrivere che l'ordine può e non deve:

Ma questo è sbagliato. Per questo abbiamo indicato che la gratuità, perché l'istituto funzioni, perché sia correttamente impostato e non sia soltanto un'enunciazione, deve valere solo per quella parte di cittadini che hanno diritto al gratuito patrocinio. In conclusione, non comprendo perché riconoscere la bontà di un istituto e poi varare una norma che ne prevede la facoltatività e non l'obbligatorietà e addirittura prefigura un eccesso. In un momento così grave per il Paese e di economia in affanno prevedere la gratuità di un istituto del genere significa non farlo varare, non farlo istituire, dalla maggior parte degli ordini. Per tutti questi motivi chiedo che siano approvati i due emendamenti che recano la mia prima firma.

Accetto la correzione; ma sottolineo che su un tema come questo un minimo di risposta da parte di chi respinge la proposta sarebbe dovuto; non per rispetto a noi, all'opposizione, ma per rispetto al Paese a cui questa legge è destinata. Ma è mai possibile che non si possa discutere con al maggioranza su un tema importante come questo? Argomenti che mi sembra siano esposti quanto meno in modo ragionevole e non ostruzionistico non debbano avere una parola di risposta da parte della maggioranza? Questo, francamente, non mi sembra un modo corretto di affrontare un tema di questa delicatezza

di astenermi da interventi che possano sembrare una replica diretta ad interventi immediatamente precedenti. Debbo però richiamare l'attenzione dei colleghi, ed in particolare del collega Ichino, sulla assoluta manifesta irragionevolezza di questo emendamento, in virtù del quale si chiederebbe tra l'altro di istituire un servizio attraverso il quale i consigli dell'ordine sarebbero, durante la fase di svolgimento del rapporto professionale, e quindi con un rapporto professionale in corso, chiamati - ad insaputa dell'avvocato che sta svolgendo la professione - a svolgere una funzione parallela di controllo circa la qualità e correttezza parallela al rapporto in corso, dovrebbe andare con le carte processuali a fare verificare ciò che l'avvocato sta facendo in quel momento in virtù di un rapporto fiduciario. Ma questa è veramente

consentire l'attivazione di un servizio gratuito di consulenza. Vorrei, allora, proporre una riformulazione anche per l'emendamento 28.203 che riguarda un tema molto importante perché parla di borse di studio per agevolare l'ingresso nella professione di giovani in situazioni di disagio economico, loro collocazione presso studi professionali, della destinazione di una parte delle risorse economiche dell'ordine. Vorrei, pertanto, inserire una clausola di questo genere: «Agli oneri derivanti dalla concessione di borse di studio, ogni consiglio dell'ordine provvederà per l'importo corrispondente ad un aumento della quota degli iscritti».

significato ideologico pregnante. Leggiamo la lettera *n)* che con questo emendamento miriamo a sopprimere: il consiglio dell'ordine «può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF». Il CNF adotta regolamenti che consentono ai consigli dell'ordine di creare dei giudici. In definitiva, di cosa si parla nel momento in cui si fa riferimento a camere arbitrali e a organismi di risoluzione alternativa delle controversie? Ad una forma di giustizia che non è privata, come negli arbitrati che sono previsti dalle disposizioni contrattuali o da disposizioni di legge, ma che non è e non può essere pubblica nel momento in cui è un organismo

da queste camere di conciliazione e da questi organismi di risoluzione alternativa delle controversie? Certamente non quella obbligatoria. Allo stesso tempo, non si può tacere il fatto che essendo organismi costituiti dal consiglio dell'ordine sarebbe possibile una pressione psicologica fortissima perché fossero adottati con una sostanziale violazione di un principio costituzionale che ha a che fare con la natura della giurisdizione. Questa norma è tecnicamente corporativa, non nel senso

del consiglio, tale organo «vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti». Non so se chi ha scritto questa norma avesse piena consapevolezza del suo significato, suo significato, perché nel gergo e nella terminologia tecnica del diritto amministrativo il potere di vigilanza è un potere specifico e pregnante, che se non allude a una sovraordinazione certamente allude a un sistema di giustapposizione amministrativa. Il consiglio dell'ordine, secondo questa norma, vigila su come vengono organizzati gli uffici giudiziari, vigila sull'attività dei magistrati. non vi è alcun dubbio che gli avvocati possano e debbano vigilare sul corretto esercizio della giurisdizione, e non nel senso tecnico e pregnante che l'espressione ha quando viene inserita in una norma che attribuisce delle competenze amministrative; ma un conto è prestare attenzione istituzionale e professionale acché le norme siano correttamente interpretate e rispettate e la giurisdizione e la sua organizzazione abbiano il migliore esito possibile, un altro è attribuire ad un ordine professionale un potere di vigilanza sull'organizzazione degli uffici giudiziari. Ripeto quindi quanto detto prima: questa è una norma tecnicamente corporativa

il Gruppo del Partito Democratico voterà contro questo articolo, perché non contiene le integrazioni che abbiamo chiesto e proposto con i nostri pochi ma precisi e puntuali emendamenti, bensì anche

al comma 1, lettera *g)*, dove si stabilisce che il Consiglio dell'Ordine esercita il controllo della continuità e effettività dell'esercizio professionale, con il conseguente potere di escludere dall'esercizio della professione i colleghi che siano ritenuti non in posizione tale da rispondere a tale requisito. Questa disposizione preoccupa gravemente preoccupa gravemente decine di migliaia di avvocati italiani che oggi vedono con vera, profonda apprensione

Data l'importanza di questa norma mi sono procurato le leggi o regolamenti che disciplinano la professione forense in Danimarca, Slovenia, Repubblica federale tedesca, Regno Unito, Spagna e Francia: non ho trovato, in queste leggi e regolamenti,

Torno a proporvi, e non solo in riferimento a questa parte della legge ma anche in riferimento a tante altre leggi che qui approviamo, adottare il criterio della comparazione come criterio fondamentale delle nostre scelte. Se in tutta Europa non esiste una norma di questo genere ci sarà pure un motivo; se siamo inseriti in un mercato europeo che è mercato comune anche dei servizi legali, percepire l'esigenza di armonizzare il nostro ordinamento rispetto alla totalità degli ordinamenti forensi in Europa, che ci consiglia di non introdurre un vincolo che graverebbe soltanto sugli avvocati italiani? A me sembra che questa sia un'esigenza elementare. Vi chiedo che di questo si tenga conto nell'emanare norme che davvero vanno contro l'interesse di gran parte degli avvocati italiani.

la settimana scorsa avevo preannunciato un'illustrazione dell'emendamento 32.202, che necessita peraltro di una precisazione tecnica, che adesso renderò. Auspico naturalmente un parere favorevole da parte del relatore e del Governo. Si tratta di una norma, messa a punto con l'aiuto di molti ordini forensi, in base nei distretti più piccoli, dove si elegge un solo delegato rappresentante nel Consiglio nazionale forense,

distretti più grandi, invece, che eleggono due rappresentanti, questo meccanismo non funzionerebbe. Allora prevedo che, nel caso in cui risulti eletto il primo in rappresentanza di un ordine circondariale, il secondo debba essere necessariamente il primo eletto di un altro ordine circondariale, non dello stesso.

io lascio inalterato il numero dei componenti; quindi non c'è variazione di spesa. Molti emendamenti tendevano ad aumentare il numero, per venire incontro a questa esigenza. Invece, in base a come ho strutturato il mio emendamento, si lascia invariato

questo provvedimento sia a carattere verticistico e che i giovani siano molto penalizzati: noi ci siamo battuti affinché si aprisse molto di più ai giovani, ma non c'è stato verso.

Presidente, un'ulteriore riflessione, attesa la delicatezza della materia, mi sembra doverosa. Pertanto, aderisco alla proposta

il nostro ordinamento costituzionale non consente di istituire un rappresentante unico ed esclusivo di una categoria professionale.

oppure tutto questo non ha alcun peso e si ritorna al sindacato unico nazionale di categoria? Credo che su questo aspetto una riflessione attenta vada fatta e che una risposta vada data. aspetto, gravemente lesiva di un principio costituzionale.

è un ulteriore tassello di quel quadro ideologico in cui si iscrivono le norme relative alla rappresentanza degli avvocati. In questo caso si parla del Consiglio nazionale forense al quale addirittura da questa norma è attribuito Il Consiglio nazionale forense è lo stesso organismo che poi deve applicare il codice deontologico ed è lo stesso organismo che nella sua qualità di giudice disciplinare dovrebbe applicare le norme che esso stesso adotta addirittura periodicamente, come in una sorta editto pretorio, essendo trascorsi però 2500. La prospettiva moderna di ridefinizione delle competenze degli organismi rappresentativi implica, in generale, un'esigenza semplice: quella della distinzione delle funzioni. Chi adotta le regole non deve essere lo stesso soggetto che le applica, soprattutto in una chiave e in una sede di tipo giurisdizionale o paragiurisdizionale. Le regole del codice deontologico dovrebbero essere adottate, e prima ancora redatte, da una commissione mista, istituita presso il Ministero di grazia e giustizia, e non già dal Consiglio nazionale forense, lo stesso organo - ripeto - che poi dovrà farle rispettare e, soprattutto, che dovrà applicare le sanzioni relative alla violazione. Voteremo, pertanto, a favore di questo emendamento e chiediamo la votazione

L'adozione del regolamento in materia di socializzazione è competenza del Ministro e non si capisce come possa essere contemporaneamente di competenza del consiglio nazionale forense. Si tratta di una norma da espungere per la ragione eminentemente tecnica che ho esposto. Voteremo,

cioè la indebita compresenza in capo ad un soggetto la cui funzione istituzionale è e dovrebbe essere quella di garantire - usando un'espressione impropria il governo e l'autogoverno della professione, una indebita interferenza in altri ambiti e, in particolare, in quello dell'amministrazione della giustizia che naturalmente è cosa che interessa moltissimo gli avvocati e sulla quale gli avvocati devono o dovrebbero esercitare il controllo più attento in tutte le sedi, ma che non può essere assegnata come facoltà e come attribuzione istituzionale ai soggetti rappresentativi della categoria. 33 attribuisce al Consiglio nazionale forense una serie di prerogative, fra queste la possibilità di esprimere, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge relativi all'amministrazione della giustizia. Non è cosa che in quanto soggetto rappresentativo della categoria degli avvocati il Consiglio nazionale forense possa fare se non a pena di una non modesta non modesta lesione di un sistema di equilibri tra poteri e competenze dei diversi soggetti istituzionali. Votiamo quindi a favore

sarebbe una indebita ingerenza da parte del Consiglio nazionale forense esprimere, e solo su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge forse non ha un fondamento preciso solo che si consideri che questi pareri su proposte e disegni di legge devono interessare congiuntamente la professione forense e l'amministrazione della giustizia. Qualche fondamento potrebbe avere ciò che è stato esposto, anche con una certa insistenza, dal senatore Carofiglio, in base al principio che una corporazione non può interessarsi dell'amministrazione della giustizia in genere,

rigetto della proposta emendativa avanzata.

Se quello che abbiamo detto prima, con sfumature, differenti posizioni e punti di vista variegati ha un minimo di senso, ipotizzare che fra le competenze istituzionali previste per legge del Consiglio nazionale forense ci sia l'istituzione di una commissione che controlla l'amministrazione della giustizia significa introdurre un elemento di grave disturbo nell'equilibrio delle prerogative dei diversi soggetti che a vario titolo in quella amministrazione intervengono. Un'indebita interferenza al di fuori al di fuori di ciò che è e dovrebbe essere attribuito all'Avvocatura, intesa come presenza diffusa di controllo su quell'amministrazione e non già come categoria che elegge un soggetto di essa esponenziale che controlla la giurisdizione.

prevede che il Consiglio nazionale forense esprima addirittura pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Che cosa vuol dire? Che cosa significa? Quali pubbliche amministrazioni? pareri al Consiglio nazionale forense da parte delle pubbliche amministrazioni? E poi per fare cosa? Per adottare provvedimenti amministrativi? Per adottare regolamenti? O perché le scelte politiche delle amministrazioni pubbliche, nella loro componente elettiva,

*(PdL)*. Mi viene il sospetto che gli argomenti resi dal senatore Carofiglio trovino una qualche condivisione nel suo Gruppo. Speravo che così non fosse, ma siccome vedo che questi emendamenti recano, oltre alla sua, anche qualche altra illustre firma, mi viene il timore che possano essere condivisi. In parole povere, con tre successivi emendamenti i colleghi presentatori pretendono che il Consiglio nazionale forense

e costituiti anche presso il Ministero non possano rendere pareri su questioni che ineriscono, non solo lo svolgimento della professione - bontà vostra (ma forse neppure ciò vorreste), ma anche il funzionamento della giustizia, su come funziona la macchina della giustizia. Ricordo che i magistrati possono farlo in tutte le sedi, essendo consulenti di tutti i Ministeri, degli uffici legislativi degli uffici legislativi dei partiti e di tutti gli organismi, considerando l'amministrazione della giustizia cosa propria. Voi,

vorreste che fossero solo i magistrati a poter disporre di tutto ciò che riguarda l'organizzazione della giurisdizione e della giustizia in senso lato e che il massimo organo rappresentativo a livello istituzionale forense non possa rendere pareri

quanto meno intimamente, da ciascuno di voi. Quindi, è un bene che siano già stati rigettati i due precedenti emendamenti, e che lo sia senz'altro anche

abbia compiti già sufficientemente gravosi per essere investito anche di una generica possibilità di esprimere i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. A me sembra che nel corpo di questa legge ciò sarebbe Sono quindi convinto delle indicazioni, non per quelle forme espresse propriamente dal senatore Carofiglio, che sono sempre molto pregnanti, ed invito il relatore e il Governo a mutare il proprio parere sull'emendamento

Per quanto vi sia una rilevanza pubblicistica del CNF (ci può stare ad esempio il parere al Ministro, se richiesto, su materie riguardanti l'amministrazione della giustizia o la professione forense

A me pare che questo eccesso di rilevanza pubblicistica vada ben oltre i limiti costituzionali e metterebbe in seria difficoltà lo stesso Consiglio nazionale forense.

pur sapendo che la norma costituzionale attribuisce al Consiglio di Stato la competenza sui pareri, debbo rimarcare che non si tratta certamente di una competenza esclusiva, quindi potrebbe ben restare, nel contesto normativo del quale ci stiamo occupando, un'ipotesi come quella contenuta alla lettera *t)*, comma 1, dell'articolo 33.

mi uniformo alle loro sollecitazioni ed esprimo parere favorevole. obiettivamente questa ulteriore funzione attribuita al Consiglio nazionale forense non aveva alcuna logica. È come se si trattasse di un parere qualificato. Il Consiglio nazionale forense svolge determinate funzioni, delicatissime e importanti, ma non possiamo attribuirgli con legge l'attribuzione di un ruolo qualificato nell'esprimere pareri qualificati. I pareri qualificati per le pubbliche amministrazioni

In dissenso dal Gruppo mi astengo, in solidarietà con la chiamata alle intime convinzioni del senatore Benedetti Valentini perché mi dispiacerebbe lasciarlo solo dopo avere contraffatto il parere del Governo e della maggioranza.

è la natura giuridica degli ordini che anche in questo provvedimento noi consegniamo al Consiglio nazionale forense come agli ordini territoriali, che è una natura giuridica di enti di diritto pubblico e quindi di enti ausiliari dello Stato. Ciò fa venire meno finanche la contestazione, l'osservazione, che in modo assolutamente argomentato ma non sufficientemente convincente ha rappresentato il senatore Ichino in relazione al comma 1 dell'articolo 33, quando si parla della rappresentanza istituzionale. La natura giuridica dell'ordine, come ente di diritto pubblico, ne fa un ente che rappresenta, nella sua funzione di ausilio allo Stato, un organo istituzionale. Da ciò discende, signora Presidente, onorevoli colleghi, una uniformità nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le attività degli ordini anche di altro tipo di professione. Tutti quanti confermano la natura giuridica e confermano anche, tra le varie funzioni, quella di esprimere i pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni. Qui abbiamo un aspetto le pubbliche amministrazioni richiedono. Non è un Consiglio nazionale forense o un ordine territoriale che spontaneamente formula un parere, la qual cosa non mi sembra neanche fuori luogo: è una pubblica amministrazione, cioè un'amministrazione dello Stato che chiede ad un ente che ha la funzione di ausilio allo Stato stesso un parere. Allora, io non sono favorevole all'abrogazione di questa lettera *t)*. Semmai aggiungerei le parole: «esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni nelle materie oggetto della competenza del Consiglio nazionale forense». Magari limiterei l'ambito del pronunziamento del parere agli stretti contenuti che hanno riferimento alla materia di competenza del Consiglio nazionale forense e degli organismi ordinistici territoriali.

mi pare che anche nella versione un po' ristretta che proponeva poco fa il collega che ha preso la parola si possa rilevare da un punto di vista strettamente formale una eccessiva dilatazione

extracostituzionale, anticostituzionale, del potere non già di parere ma di veto. Ormai ci sono volumi e volumi di colleghi di diritto costituzionale che parlano del Consiglio superiore della magistratura, neanche come terza Camera, ma come seconda e dove la prima è «Porta a Porta», la Camera ed il Senato vengono dopo. Allora, se questo profilo non ci deve sfuggire, non possiamo ragionare nei termini pur corretti dal punto di vista della legislazione ordinaria che ci ha richiamato nel merito il collega Centaro. Quindi, mi sento di invitare il relatore ad una formula che tenga presente i sentimenti e gli argomenti espressi da Benedetti Valentini e sulle quali ho visto vi è una rispondenza da parte anche di colleghi di questa parte. Altrimenti noi stiamo in un dibattito un dibattito che sembra veramente isterilito tra combattenti e reduci dell'associazione nazionale magistrati, in questo caso la prima volta non vi è stato l'intervento liberistico del collega Ichino con la solita citazione di Alessandro De Nicola su

Libertà: una libertà di opinioni come questa non si è mai ricordata ma non è un gran merito in questo caso perché l'emendamento è di così modesta portata, ove lo approviamo o lo bocciamo. L'importante è che siano stati bocciati i due precedenti. Quindi non è poi così importante. Mi limito a dire, anche se certamente la mia dottrina non merita l'aggettivo di illustre perché è umilissima, anzi addirittura oscura, che non vedo che non vedo come si possa non concepire che un'importante amministrazione pubblica - che so - un grande Ente previdenziale od altro non possa richiedere al Consiglio nazionale forense - che so un parere su una bozza di convenzione per la stipula dell'assistenza legale sul territorio nazionale o quant'altro, così come lo farebbe localmente con gli ordini territoriali. È assolutamente inconcepibile. Quindi, restando umilissimamente e senza dottrina del mio parere,

favorevole su

preselettiva di accesso al tirocinio. Non solo lo regolamentiamo diversamente, ma vogliamo soprattutto sopprimere una prova che non trova nessuna giustificazione.

emendamenti che riguardano il comma 12 dell'articolo 39, che il praticante possa chiedere di cambiare lo studio presso cui svolgere il tirocinio; invece che essere autorizzato dal Consiglio Consiglio dell'Ordine, che valuta e notifica, si chiede cioè che il Consiglio dell'Ordine prenda atto di tale decisione del tirocinante che chiede di cambiare studio professionale.

potrebbe essere logico che chi fa pratica non possa avere un impiego a tempo indeterminato, un impiego fisso presso una pubblica amministrazione; ma che si escluda per chi vuol fare la pratica e quindi cercare di fare l'avvocato qualunque rapporto di impiego pubblico mi sembra francamente incongruo e irragionevole, perché ciò esclude un rapporto di collaborazione, quindi parziale, esclude ad esempio un rapporto serale, che potrebbe essere un impiego presso È un'esclusione che mi sembra ingiustificata e estremamente penalizzante per chi può far pratica ma, al tempo stesso, avere un qualche forma di collaborazione e di rapporto di impiego pubblico, anche parziale e provvisorio. Mi sembra una penalizzazione davvero incomprensibile. Certo, poi è prevista l'incompatibilità con l'impiego pubblico per chi diventa avvocato, ma nella fase di praticantato mi sembra davvero una norma che andrebbe corretta oppure ridotta. Pensiamo alla collaborazione di un avvocato non può far pratica e fornire una qualche collaborazione, una qualche consulenza? Credo che su questo divieto così perentorio vada fatta una riflessione per arrivare, se possibile, ad un ripensamento.

Dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-*bis*. I costi per la costituzione e il funzionamento delle commissioni, nonché per l'espletamento della prova di ingresso devono essere a carico dei singoli consigli dell'ordine». **39.215**

Signora Presidente, il fatto che abbiamo già all'ordine del giorno, domani alle ore 19, la presenza del Governo per parlare delle alluvioni che hanno toccato il Veneto ed altre parti d'Italia mi rassicura. Tuttavia mercoledì scorso, in questa sede, avevamo chiesto che il Governo, oltre a raccontarci i fatti, venisse già con il preventivo. è tenuto un Consiglio dei ministri che ci ha profondamente deluso. Oggi si sono impegnati il presidente Berlusconi ed il ministro Bossi.

e finanziamenti - perché i nostri sindaci e le nostre popolazioni hanno un tale livello di dolore e di sofferenza che stanno davvero sfiduciando le istituzioni. Noi, da questo luogo, dobbiamo recuperare la loro fiducia. Si aspettano la solidarietà di tutta l'Italia e credo che noi siamo nelle condizioni di darla a tutto il Paese: al Veneto, alla Liguria, alla Toscana a tutti quei cittadini che pensano che questa sia la sede nella quale il Governo, confrontandosi, può scegliere le priorità e quindi anche stabilire gli stanziamenti dovut**i.** *(Applausi del

sembra davvero singolare e irrispettoso anche della forza politica che usa quello stesso simbolo. Se io faccio parte di una forza, nel momento in cui vengo eletto sindaco rappresento tutti i cittadini: sarebbero guai se non fosse così!

Signora Presidente, mi corre l'obbligo di intervenire nel tentativo di chiarire meglio alcune informazioni che sono state poc'anzi fornite dalla senatrice Mariapia Garavaglia nel suo intervento. Le condizioni del nostro Veneto sono note a tutti, anche a chi magari non ha, come noi, la ventura di vivere in quei territori. Quindi, non mi dilungo oltre sull'entità dei danni che è davvero cospicua. l'obbligo di ricordare alla senatrice Garavaglia che il Veneto non è stato e non sarà lasciato solo dal Governo nazionale;

stanno dimostrando l'assoluta vicinanza delle istituzioni. Non c'è nessun Veneto che si sente lontano dalle istituzioni: è rappresentato dalle proprie istituzioni regionali e nazionali. nella consapevolezza che il territorio del Veneto versa ogni anno allo Stato 12 miliardi di euro attraverso la propria tassazione, crediamo possa essere assolutamente condivisibile la proposta che sale dai territori veneti di vedere riconosciuto l'aiuto ed il sostegno in questa fase di grande difficoltà per le famiglie e le nostre imprese. Siamo certi,

alla ricostruzione del tessuto produttivo sarà garantito dall'Unione europea. Raramente il buon funzionamento delle istituzioni si si è dimostrato possibile come in questa occasione. I sindaci di quei Comuni lo sanno bene e incontreranno l'11 novembre prossimo il Presidente della Repubblica

stata di estrema importanza, significativa, efficace ed efficiente. Siamo sicuri che questa triste pagina della storia veneta, determinata da questa alluvione, potrà concludersi

Signora Presidente, l'intervento della senatrice Baio ci impone una brevissima replica. Infatti, quando le istituzioni statali sentono addirittura il dovere di intervenire sul gonfalone di un Comune e sulle decisioni che un sindaco ed una comunità